6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Nella seduta di ieri pomeriggio

un rinvio in Commissione del provvedimento riguardante il codice antimafia. Io credo che l'inizio di questa seduta sia

molti Presidenti emeriti della Corte costituzionale si siano espressi chiaramente dicendo che il provvedimento è incostituzionale e il fatto che il presidente dell'Autorità anticorruzione,

sua decisione, evidenziando il fatto che delle novità sono accadute. Nel caso la sua decisione fosse negativa, ossia se il suo giudizio, che in questo caso è insindacabile, fosse diverso dal mio (cosa non soltanto legittima, ma assolutamente possibile), allora le chiederei un'inversione dell'ordine dei lavori, che è invece nelle facoltà

propone alla Camera di prendere in considerazione le osservazioni del presidente Cantone di procedere a una revisione del disegno

il testo non è controverso per la restante parte - e cioè l'introduzione di taluni delitti contro la pubblica amministrazione nel novero di quel titolo di reati che consente l'applicazione delle misure di prevenzione. prevenzione. Dobbiamo fare una premessa, perché non è pensabile che la verità sia divenuta un fatto del tutto irrilevante. Il Senato per primo - e unicamente - ha posto il problema in questa direzione; tant'è che noi abbiamo scritto un testo alternativo, interno alla Commissione, nel quale certamente i delitti contro la pubblica amministrazione non compaiono tra i delitti che possono attivarne l'applicazione.

quanto alle misure di prevenzione. Quindi, il Senato ha trovato una soluzione, essendo stato l'unico ramo del Parlamento che si è posto il problema. Noto, con dati oggettivi di fatto e con date, che il testo viene introdotto alla Camera dei deputati nel novembre 2013, vi rimane sino al 2015 e, all'interno dei lavori della Camera dei deputati, si verifica la introduzione delle disposizioni cosiddette incriminate. Devo rilevare che nessuno ha sollevato il problema. Ciò avviene in un contesto di assoluto silenzio, di acquiescenza e - in un certo senso Il Senato pone il problema. Lo risolve in una maniera che io posso pensare, astrattamente, possa a taluno anche non piacere. È un problema di natura giuridica, che la Camera dei deputati potrà potrà eventualmente risolvere. Ma è paradossale che il problema esploda all'interno del Senato, unico ramo del Parlamento che sottolinea la difficoltà di una scelta legislativa e lo fa all'interno del proprio dibattito. Basterebbe, una volta tanto, per amore della verità, andare a leggere i Resoconti del Senato, dai quali risulta, in maniera chiara, che il Senato quella soluzione non apprezzava e, intanto, per una ragione che va detta:

alle soluzioni che si diedero con il pacchetto sicurezza del 2008-2009. Certo, nel passare da un sistema di reiterazione a un sistema in virtù del quale bastava un unico reato per determinare l'applicazione delle misure di prevenzione al Senato, quando nessuno aveva posto il problema, quando - anzi - la stampa spingeva in questa direzione, affermando, con articoli che turbano i lavori parlamentari, che quelle perplessità significavano voler sottrarre i corrotti alle misure di prevenzione, è inevitabile che guasti di siffatto genere si determinino. Comunque, io devo dare una risposta alle richieste.

si sottometterà a qualsiasi decisione dell'Assemblea. Noi riteniamo, però, improponibile il rientro in Commissione di un testo approvato dall'Assemblea. Qui rimane soltanto, per ragioni puramente formali, di ordine e organizzazione dei lavori, l'approvazione di un ultimo articolo. La Camera dei deputati, che questo problema, a a torto o a ragione, ha determinato attraverso l'introduzione di una disposizione che il Senato e, soprattutto, la Commissione giustizia non hanno apprezzato sin dal primo momento, potrà fare questa correzione e, e, conseguentemente, sarà poi il Senato valutarne la condivisibilità. Ma in questa fase è del tutto impensabile che il testo rientri in Commissione. Lo dico con molto rispetto: nessuno pensi che questo aggettivo sia

in parte anche su quella del senatore Caliendo, innanzitutto, per quanto riguarda l'inversione dell'ordine del giorno, devo rilevare che siamo già entrati nell'ordine del giorno. Quindi, è impossibile procedere all'inversione. E questa era la subordinata proposta dal senatore Quagliariello. Per quanto riguarda l'istanza correttamente qualificata come questione sospensiva tardiva per fatti nuovi sopravvenuti, con una valutazione

Signor Presidente, soltanto per assoluta trasparenza e per

per quale motivo, essendosi aperta la seduta con un ordine del giorno, tale ordine del giorno non possa essere invertito. Io ritenevo, e forse sbagliando, che una tale richiesta potesse intervenire in qualsiasi momento da parte di un senatore.

Intanto chiarisco che, avendo detto «passiamo all'esame dell'articolo» e avendo poi dato a lei la parola, abbiamo già iniziato la trattazione dell'ordine del giorno.

venga proposto e illustrato da soggetto diverso, ancorché autorevole, come il presidente Cantone, non rappresenta alcuna novità. Personalmente ritengo che molte voci in quest'Aula,

quando parla il presidente Cantone, vedono, eventualmente, un fatto nuovo in ciò che è indubbiamente vecchio. Ho grande considerazione e ammirazione per il presidente Cantone ma, se vuole, può venire qui a prendere il posto di tutti noi e fare le leggi, lasciando l'autorevolissimo e prestigiosissimo incarico che ricopre. Io dico che

Faccio riferimento all'intervento del collega Falanga. Non avevo ritenuto che il fatto nuovo fosse soltanto

come ha evidenziato l'Unione delle camere penali, sia sul fronte dell'efficacia della repressione del crimine. Il codice antimafia che stiamo discutendo è riuscito in questo miracolo. Signor Presidente, colleghi, se abbiamo fatto riferimento in particolare all'intervento del presidente Cantone e ai rilievi critici del procuratore Roberti è perché riteniamo che il loro ruolo sia istituzionale e debba essere tenuto presente proprio perché è istituzionale.

tirato in ballo troppo spesso. Addirittura un giorno lessi una sua intervista sul «Corriere dello Sport»: sembrava essere diventato l'allenatore del Napoli, cosa che mi preoccupò innanzitutto come tifoso e poi anche come senatore. In questo caso, invece, i suoi giudizi hanno un rilievo importante per il ruolo istituzionale che Cantone ricopre, così come i giudizi di Roberti hanno un rilievo particolare per il ruolo istituzionale che egli riveste. Devo dire, signor Presidente, che mi ha molto colpito il fatto il presidente D'Ascola abbia detto che il dibattito in Commissione è stato molto ampio e che le audizioni non sono mancate, ma non è normale che nessuno abbia pensato di

beneficio del collega Falanga, che oltre a Cantone sono intervenuti moltissimi altri giuristi e, soprattutto, molti Presidenti emeriti della Corte costituzionale. Flick segnala che, facendo confusione tra sanzione e prevenzione (con quella che Luciano Violante, anche lui ferocemente critico nei confronti di questo testo, ha chiamato con efficacia "truffa delle etichette") *(Commenti a mettere in confusione persino la Corte di Strasburgo. Il presidente Flick ci spiega che finora le corti sovranazionali si sono trovate a giudicare strumenti eccezionali pensati per contrastare fenomeni eccezionali, come quello della criminalità mafiosa: estenderli all'ordinario significa che, prima o poi, potrebbe arrivare da Strasburgo una pronuncia che metta in discussione lo strumento in sé. Il tema ha peraltro aspetti paradossali. Come infatti segnala il neoprocuratore della Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, a lungo pubblico ministero della Procura nazionale antimafia, signor Presidente, e come parimenti ci spiega Giovanni Fiandaca, l'attuale sistema di prevenzione funziona già oggi non solo per i mafiosi, ma anche per i corrotti e i grandi evasori. Dobbiamo essere consapevoli che le modifiche di cui stiamo discutendo in Senato rischiano di mettere a repentaglio l'utilizzo dello strumento. Il rischio di incostituzionalità e di incompatibilità con le convenzioni internazionali è segnalato anche da Cesare Mirabelli e da Giuseppe Tesauro, Presidenti emeriti della Consulta, e da Sabino Cassese, ex giudice costituzionale: tutti avvertono rispetto al rischio che l'illegittima estensione all'ordinario di uno strumento straordinario, come quello della prevenzione, delegittimi l'uso stesso dello strumento, arrecando un danno irreparabile alla lotta alla criminalità organizzata. In questo quadro appare quasi mite il giudizio del solitamente graffiante di Carlo Nordio, secondo il quale questa norma «non servirà assolutamente a nulla», come le tante norme segnaletiche che in questi anni - spiega - hanno «aumentato la confusione e ridotto le garanzie senza intimidire i corrotti». Come vede, signor Presidente, e come può notare anche il collega Falanga, non è soltanto il giudizio di Cantone ad essere stato preso in considerazione: si tratta di un concerto, al quale hanno partecipato Presidenti emeriti della Corte costituzionale e responsabili di importanti istituzioni. Mi rifaccio alle giuste considerazioni del collega Caliendo: nel momento in cui viene già annunziato un intervento dell'altro ramo del Parlamento, in prossimità della fine della legislatura, chiedo in particolare ai colleghi del Partito Democratico se non sia più saggio provare a correggere qui il provvedimento, in modo tale che la Camera dei deputati possa poi approvarlo e che non vi sia bisogno di due letture. Questo, signor Presidente, non perché una lettura in più sia uno scandalo, come lei tante volte ha segnalato, ma perché, tenuto conto del momento della legislatura in cui il provvedimento viene a cadere, sarebbe possibile che non si arrivi in porto. Credo che, in questo caso, un supplemento di responsabilità potrebbe evitare tale esito. In questo senso chiedo nuovamente il ritorno in Commissione del provvedimento,

Lei non può. Ho posto in votazione la sospensiva richiesta dal senatore Quagliariello.

*(FI-PdL XVII)*. Sì, ha parlato prima. Ma il senatore Caliendo ha parlato di un'altra cosa. Sulla proposta del senatore Quagliariello non c'è stato un intervento del Gruppo di Forza Italia. Quindi la prego di dare la parola al senatore Malan, perché si possa esprimere su questa proposta.

un commentatorio. Questo è il Senato della Repubblica, di cui lei è la prestigiosa figura di vertice che lo rappresenta e deve far rispettare il Regolamento, il quale stabilisce che sulla proposta del senatore Caliendo, che lei ha ammesso,

dal dottor Cantone, ma quanto affermato in seguito dal Presidente del Partito Democratico (che ha la maggioranza relativa sia al Senato, che alla Camera

In ogni caso, anche qualora venga richiesto il sostegno per la votazione a scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trattandosi dell'unico emendamento presentato, si procederà al voto sul mantenimento dell'articolo 36.

Sull'articolo 36, oltre all'emendamento presentato dal senatore Caliendo, c'è

Ho capito, ma sta parlando il senatore Azzollini, che ha posto un problema e io ho chiarito il punto della discussione. Siamo sull'emendamento Siamo sull'emendamento 36.100. Senatore Azzollini, concluda il suo intervento.

il mantenimento dell'articolo 36 avrà la possibilità di parlare. La votazione della proposta di coordinamento sarà successiva.

Poiché l'articolo 36, quale che sia l'esito dell'emendamento Caliendo, verrà poi posto in votazione, si potrà sostenere più tardi che non si possa intervenire sull'articolo 36 perché lo avremo già votato. Invece, su quell'articolo voglio parlare perché nella proposta di coordinamento, che lei mi dice successiva, si parla dell'articolo 36. Non mi voglio trovare di fronte a una preclusione; pertanto, le chiedo di dirmi quando posso parlare ampiamente sulla questione di copertura di cui all'articolo 36. Se vuole parlare sull'articolo 36, può farlo adesso. Se vuole parlare sulla proposta di coordinamento, può intervenire successivamente, però noi dobbiamo procedere, secondo il Regolamento, alla votazione sul mantenimento dell'articolo. Se vuole parlare sull'articolo 36,

richiamo al Regolamento, perché, come sicuramente ricorderà, il comma 9 dell'articolo 100 recita «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo» - l'emendamento è presente perché soppressivo, anche se poi voteremo il mantenimento dell'articolo stesso - «si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti». Questo certifica che ciascun senatore, anche se non presentatore di emendamenti, può intervenire sull'articolo, quindi non solo uno per Gruppo. PRESIDENTE. Nessuno ha messo in dubbio questo, senatore Calderoli, né ha precluso

Ho chiesto la votazione per parti separate, sopprimendo quella parte in Commissione, e vi è stato il voto contrario. Poi vi è stata una modifica in Aula. Signor Presidente,

tant'è vero che dice che si tratta di una cosa che la giurisprudenza ha già fatto, solo che non ha capito che il mio emendamento non è stato approvato, altrimenti tutto avrebbe coerenza nel suo intervento.

dai relatori, ma mantenendo la stessa logica: al comma 4, infatti, vi è una spesa ulteriore per quanto concerne le dieci unità che possono essere assunte per il 2018 a tempo determinato.

gli stessi relatori oggi presentano un altra proposta di coordinamento, in cui dicono che all'articolo 27 della legge

tutti vengono pagati con i soldi che saranno attribuiti all'Agenzia dalle amministrazioni di provenienza. Tuttavia, signor Presidente, il trattamento accessorio relativo a queste persone

perché noi stiamo assistendo a un procedimento legislativo viziato in tutto e per tutto. Abbiamo fatto dei coordinamenti che non hanno avuto la possibilità di essere emendati,

se vogliamo definirlo in maniera corretta vorrei dire - e mi rivolgo anche alla senatrice Bianconi che ha accusato i senatori della Commissione giustizia e il Senato di essersi accorti all'ultimo momento di questi problemi che il 26 aprile 2017, in Commissione giustizia, i senatori Caliendo e Giovanardi hanno chiesto la soppressione dell'articolo 1, chiedendo cosa c'entrasse la lotta alla corruzione con la lotta alla mafia, estendendo - come è stato fatto - tutta la strumentazione delle confische dai reati antimafia a tutti quelli della pubblica amministrazione. Abbiamo sollevato quindi il problema,

sulla lotta alla mafia (come detto ieri), fa pensare a menti raffinatissime che vogliono travolgere la legislazione antimafia attraverso un meccanismo di allargamento che non ha alcun senso. quindi davvero in pericolo la lotta alla mafia e gli avvertimenti che vengono da autorevoli personaggi vanno proprio in questa direzione: voi rischiate di travolgere una strumentazione che ha passato il vaglio della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e anche dell'Europa perché, estendendola anche a singoli reati associativi, senza alcuno dei presupposti richiesti dalla lotta alla mafia, rischiate di far cadere l'intero armamentario. Mi associo quindi alle parole del senatore A proposito di ostruzionismo, ricordo che sul resto del provvedimento, in materia di lotta alla mafia, c'è il consenso di tutto il Parlamento. Questa è la cosa incredibile. Potrebbe essere licenziato un provvedimento

Su un aspetto che non ha né capo né coda, come la questione della corruzione inserita in maniera maldestra, denunciata fin da aprile e che si è tentato di correggere con emendamenti sui quali la maggioranza, facendo ostruzionismo contro se stessa, arriva addirittura a dire che alla Camera lo modificherà. modificherà. Se perdiamo qualche minuto è per cercare di convincervi di una follia che, dal punto di vista razionale, non ha né capo né coda. coda. Si tratta semplicemente di correggere le cose che assolutamente non vanno e di farlo senza dire che ce ne siamo accorti solo all'ultimo secondo, perché sono tre mesi che ce ne siamo accorti; il problema è che non se ne è accorta la maggioranza.

della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Scelgo, a caso, due commi che smentiscono platealmente questo assunto. Per la delega, di cui all'articolo 32, «si provvede», provvede», dice il testo della legge, «nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» e indica anche le fonti di copertura. Questo significa che, mentre il

Signor Presidente, non è possibile che lei ammetta questo

effetto immediato.

proposte di coordinamento: il Presidente può solamente regolare il dibattito e poi porre in votazione le varie proposte. Non può rispondere alle domande a cui devono rispondere i relatori ed il Governo.

I problemi vanno posti ai relatori ed al Governo e non al Presidente, che non ha il potere di eliminare quello che è stato proposto.

Il coordinamento, signor Presidente, è qualcosa che attiene a una migliore definizione

me stesso e anche come sussidio ai relatori quanto prevede l'articolo 103 del Regolamento: «prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte». signor Presidente, è evidente che una proposta di coordinamento non trova corrispondenza con quanto scritto sul foglio distribuito. Infatti, quanto previsto dall'articolo 36, contenuto nella proposta di coordinamento, costituisce un vero e proprio emendamento:

la proposta di legge e gli emendamenti e accorgersi che all'articolo 27 corrisponde esattamente una proposta di spesa, prevista nel provvedimento stesso. provvedimento stesso. Questa proposta di coordinamento ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio emendamento, come dicevo. «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32» significa che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Capisco che i relatori possano essere distratti e, pascolando in giro per l'emiciclo, non si ritrovino più nel provvedimento, perché ormai ne hanno perso il senso; ma il Presidente della Commissione bilancio, sempre tanto puntuale e attento, che dimostra anche disponibilità,

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32"». Noi voteremmo, come emendamento, prima dell'articolo 36, questa

Signor Presidente, io non sono d'accordo sul fatto che si tratti di una modifica sostanziale. per la semplice ragione che si tratta di una precisazione che armonizza il testo,

nell'articolo 32. Questo inciso è semplicemente una formulazione che evita equivoci interpretativi rispetto al testo, perché la previsione di spesa è già nei due commi. Quindi, non è una modifica sostanziale ma una tipica norma di coordinamento che, per evitare che il provvedimento abbia una contraddizione interna,

L'articolo 36 è la norma finale di chiusura sulla mancanza di spese; perché non vi sia contraddizione con quanto detto prima, si precisa questo fatto con un coordinamento, con un inciso che raccorda il testo nel suo complesso. Non è una modifica sostanziale.

pone un problema regolamentare, e allora il nostro Regolamento deve essere rispettato, oppure non lo pone. Ma non si può dire ai colleghi: «Se non ne approfittate, allora rispettiamo il Regolamento, altrimenti ce lo mettiamo sotto i piedi». Dico questo anche *pro futuro*. L'intervento voleva significare proprio

voglio ribadire al senatore Quagliariello che la mia è la posizione di chi ritiene che quell'inciso non sia una modifica sostanziale perché è semplicemente un coordinamento del testo nel suo complesso per evitare, alla luce dei criteri di interpretazione, che possa sorgere un dubbio nel momento in cui si va ad interpretare il testo. Quell'inciso, dal punto di vista normativo, nulla a ciò che è già stato votato ed è semplicemente un richiamo al fatto che, stante l'invarianza complessiva del provvedimento, esso contiene due disposizioni che prevedono spese. Questa non è una modifica sostanziale

io non ne faccio una questione di impossibilità di dialogo ma questa è la mia posizione. interpretazioni come quella del senatore Quagliariello, lo ribadisco: la mia posizione è questa e non sono disponibile a trasformare la proposta in emendamento.

però, non è un contrasto di merito, bensì è relativo ad una copertura. Non si può dire: «Questo provvedimento non porta maggiori oneri per le finanze pubbliche tranne per i punti in cui si spende». Sarebbe una presa in giro

Presidente, mi consenta una piccola annotazione che vuole essere un suggerimento assolutamente non polemico: il senatore Pagliari, oltre ad essere un senatore, è anche un buon avvocato quindi

il dibattito diventa confuso e si cominciano a difendere le proprie la più antica e famosa definizione di sostanza, talché una cosa è sostanziale e non formale: la sostanza è l'essenza necessaria di una cosa, ciò che fa sì che una cosa sia quella che è e non sia un'altra cosa. cosa. Se invece di Aristotele volessimo ricordare un filosofo del diritto più vicino il senatore Ceccanti, nel suo testo di diritto parlamentare, ricorda che il coordinamento, che avviene dopo le dichiarazioni di voto prima del voto finale, ha il significato di coordinamento formale. di modificare la portata dell'articolo 36, è indubbio (quindi stiamo parlando di una cosa che non esiste) che la portata sia sostanziale e non formale. Presidente, lei è enormemente rispettoso

ulteriori problemi, di agevolare i relatori. Se la preoccupazione è quella di possibili

chiedere ai relatori di presentare l'emendamento (in caso diverso, dovrebbe prendere ulteriori decisioni) e porre fine a questa discussione. Si tratta di una discussione anche spiacevole, perché perché porta lei a dover gestire una situazione difficile, porta agli estremi il dibattito in Aula e, se mi permette, potrebbe in futuro determinare anche una certa disponibilità dei critici, che sono notevoli nei confronti del Parlamento, a dire che ci interessiamo ci interessiamo di questioni a questo punto soltanto formali e procedurali, ancorché sostanziali. Le rinnovo la proposta: ponga fine alla discussione e inviti

Presidente, sembra quasi che ogni volta che chiedo di parlare vi sia distrazione, il mio intervento possa essere contrario a qualcuno. Nel caso di specie, Presidente, devo dire la verità, la mia posizione è assolutamente identica a quella che mi sembra essere la sua. Non riesco davvero a comprendere quello che sta accadendo. Abbiamo un problema sull'articolo 36

le perplessità che le sono state rappresentate in quest'Aula circa la natura del coordinamento formale proposto dai relatori. Tanto ciò è vero che, ripetutamente, ha invitato i relatori - così mi è parso di comprendere - ad assumere un'iniziativa diversa. adesso ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo, perché quando il relatore Pagliari dice che egli la vede così e non è assolutamente disponibile a cambiare idea e a presentare un emendamento, signor Presidente, a quel punto deve intervenire. Infatti, nel momento in cui lei condivida le perplessità che abbiamo sulla natura di coordinamento formale, non possiamo più andare avanti, a meno che, evidentemente, i relatori non si convincano della trasformazione di quella proposta di coordinamento formale in un emendamento. Dico di più, signor Presidente:

- ma siamo un'istituzione e abbiamo necessità di prudenza e di moderazione. Siccome stiamo ultimando il procedimento legislativo con riferimento ad un disegno di legge di estrema delicatezza, prudenza vorrebbe, a fronte dei dubbi seri che sono stati esposti, che si presenti un emendamento, sul quale si pronuncerà la Commissione bilancio.

non di impuntarsi sulle proprie idee. Concludendo, signor Presidente, siccome ritengo che la Presidenza eserciti un ruolo molto diverso da quello del distributore di minuti, credo che un suo autorevole intervento possa far superare questa situazione di stallo. Dunque le chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti, non di più:

ha fatto capire che con il coordinamento, che è un fatto tecnico finale, non si può risolvere un problema di sostanza, che richiede un emendamento. Pertanto, credo che il relatore, ostinandosi in questo modo,

Signor Presidente, è vero che in questa fase gli emendamenti possono essere presentati dal Governo o dal relatore, tuttavia l'articolo 100 del Regolamento, al comma 5, afferma che «il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti» in casi come quello al nostro esame. Siccome il Presidente - mi consenta di dirlo - ha rivolto un invito ad emendare, perché ha fatto capire ai colleghi che la situazione non si può risolvere con il coordinamento del testo, se da qui a mezz'ora pensate

la Commissione bilancio è stata chiamata in causa da diversi colleghi e adesso anche da lei. Ora, dal punto di vista della Commissione bilancio, quello che rileva è che i due articoli, come emendati, che comportano oneri sono stati approvati regolarmente, quindi hanno avuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, perché gli oneri sono stati quantificati e coperti. Quindi ha ragione il senatore Pagliari quando dice che dal punto di vista sostanziale tutto è a posto. C'è tuttavia un problema evidente, cioè l'imbarazzo dell'Assemblea di dover votare adesso un articolo 36

imbarazzo procedurale, perché questo articolo 36 sarà perfetto solo nel momento in cui verrà approvata la norma di coordinamento. Dopodiché, qui il Presidente della Commissione bilancio, che già è accusato di debordare - anche grazie alla mole - rispetto alle sue competenze, si ferma, perché si tratta di una questione che riguarda la procedura d'Aula.

Dopodiché, come questa condizione debba essere sanata, se con un emendamento previo o con un voto successivo, l'importante è che alla fine il testo sia così.

dal punto di vista formale c'è un imbarazzo procedurale, dal quale credo si possa uscire con un po' di buonsenso da parte di tutti, quello cui il Presidente ha richiamato l'Aula. ringrazio, presidente Tonini, per la chiarificazione di questi temi e anche per la disponibilità eventualmente a un emendamento da parte della Commissione bilancio, considerato

in relazione esclusivamente a quanto ha detto il senatore Tonini, accettiamo di presentare l'emendamento.

Vorrei chiarire che, essendo un emendamento ammesso *ex* articolo 100 da parte del Presidente, che lo ritiene assolutamente necessario, i subemendamenti non ci dovrebbero essere, quindi non sono ammissibili.

È un emendamento presentato per soddisfare un'esigenza di bilancio che è stata rappresentata lodevolmente da tutti e che si può risolvere in

Presidente, sto parlando. Mi consenta di finire senza interruzioni.

Abbiamo risolto un problema gravissimo.

così. Io ho però rilevato che quell'articolo, così come scritto, non è conforme alla volontà della Commissione bilancio.

«Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia». Costituzione doveva essere soppresso questo comma. Il comma è stato riscritto con un emendamento di coordinamento per l'Aula dai relatori e vi prego di leggerlo, perché è la stessa cosa: «Il Direttore dell'agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti

perché, altrimenti, veramente ci prendiamo in giro: utilizziamo l'articolo 81 per poter giocare a seconda delle convenienze. lei ha anticipato che, nel caso venisse presentato un emendamento dai relatori, non avrebbe concesso il termine per i subemendamenti. Io, per la verità, sfogliando il Regolamento, questa previsione non l'ho rinvenuta. Ella ha precisato che, trattandosi di un emendamento necessario, non si concedeva il termine per i subemendamenti.

Se è una sua valutazione sull'incisività e l'importanza dell'emendamento dei relatori, va bene, ma non basta e credo che non sia sufficiente per impedire a noi di esercitare il nostro ruolo e eventualmente di subemendare ciò che

Se è relativo esclusivamente all'esclusione degli articoli 27 e 32 rispetto alla non onerosità della legge, allora l'emendamento è obbligatorio e non è subemendabile.

Innanzitutto, voglio chiedere alla Presidenza o al relatore se, allo stato della discussione, il comma 4 sia rimasto identico a quello che leggiamo nell'allegato A,

- non può essere votato così com'è, per evidente contraddittorietà con l'articolo 81. Prima dico perché, poi cito la fonte e lo chiedo anche al Presidente della Commissione bilancio. Come vedete, lì manca l'annualità dell'onere. Si dice che c'è un onere di 20 milioni per il

ammortizzatori sociali, specificando se i 20 milioni di euro a carico del fondo occupazione, previsti per la copertura degli stessi ammortizzatori, si riferissero complessivamente al triennio e in tal caso occorreva indicare l'importo annuale,

il ragioniere generale dello Stato (in questo caso la relazione tecnica era firmata proprio la lui) già osservava questo punto. C'è, signor Presidente, quello che mi pare si chiami *argumentum a contrariis*: lo dico con molta modestia, perché lei sa che non mi occupo di

ottenere la valutazione della Commissione bilancio, perché dobbiamo capire se l'onere è di 60 milioni, cioè 20 per anno, o

Devo invece riconoscere che questa obiezione è fondata e che, così come è formulata, la norma di copertura non va bene; vi è quindi bisogno di un supplemento di analisi.

Questa parte del provvedimento va riportata in Commissione e i relatori devono portare un emendamento che specifichi l'entità dell'onere o la

È un dubbio che non può essere lasciato. Convochiamo la Commissione perché c'è bisogno anche dell'apporto del Governo rispetto a questo tema: trattandosi di stanziamento di risorse, il problema non

4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». Mi corre l'obbligo di precisare, signor Presidente, che la Commissione ha preso atto di questa proposta del Governo ma i Gruppi delle opposizioni hanno chiesto che tale proposta del Governo fosse corredata di relazione tecnica bollinata dal Ragioniere questo richiede un po' di tempo. Per le ore 14,30, quando la Commissione è riconvocata, disporremo di questa relazione tecnica, almeno così si è impegnato a fare il vice ministro Morando, che era presente a nome del MEF. Dopodiché, non posso che rimettere a lei e alla Presidenza l'*iter* procedurale. Sono anche incerto nel capire in che misura noi possiamo votare e cosa esattamente stiamo votando in Commissione bilancio.

attesa dell'esito di questo ulteriore completamento dell'*iter* dal punto di vista tecnico. Dopo decideremo la procedura da seguire.